Signor Presidente, considerata l'analogia dell'argomento trattato rispondo, come annunciato, congiuntamente alle interrogazioni del senatore Lombardo. La presenza invasiva del granchio blu nei mari antistanti le coste nazionali merita particolare attenzione, in considerazione del fatto che l'anomala proliferazione di questa specie aliena comporta danni gravi ai prodotti della *molluschicoltura**,* atteso che trattasi di una specie che non ha predatori naturali. Per tali ragioni, il Ministero ha immediatamente attivato, a valere sui fondi nazionali, misure di sostegno in favore delle imprese colpite che hanno provveduto alla cattura e allo smaltimento della predetta specie. Nello specifico, al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu e di impedire l'aggravamento dei danni determinatesi, a far data dal 1° agosto 2023 l'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2023 ha autorizzato la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura e allo smaltimento della già menzionata specie. Le istanze pervenute sono state tutte liquidate entro il dicembre 2023. Inoltre, al fine di dare continuità agli interventi a supporto del settore ittico e contenere gli effetti della crisi economica generata dalla prolificazione della specie granchio blu, con decreto del 13 novembre 2023 il Ministero ha destinato 10 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per sostenere una rapida ripresa del settore, indennizzando le imprese per la semina, il ripopolamento e la protezione e la protezione degli allevamenti. Il provvedimento ha previsto il rimborso delle spese sostenute per il prodotto immesso già nell'anno 2022, nonché per l'acquisto di strutture fisse e mobili istallate per la protezione degli allevamenti nell'anno 2023. Sempre in tale ottica, ricordo che con la legge finanziaria 2024 è stato modificato il decreto legislativo n. 102 del 2004 ed estesa conseguentemente l'operatività del Fondo di solidarietà nazionale anche alle imprese e ai consorzi dell'acquacoltura e della pesca. A seguito della modifica legislativa, al fine di riattivare le misure in questione, sono stati predisposti due provvedimenti ministeriali notificati quali aiuti di Stato in esenzione, ai sensi del Regolamento UE 2022/2473. 2022/2473. Ciò posto, mi preme evidenziare che lo scorso mese di agosto è stato nominato quale Commissario straordinario per l'emergenza granchio blu il dottor Enrico Caterino, ex prefetto di Ravenna. La nomina del Commissario per elaborare una strategia e uscire dall'emergenza granchio blu evidenzia la determinazione del ministro Lollobrigida e di tutto il Governo nell'affrontare il problema in maniera risoluta. Al riguardo, rilevo che, per l'attuazione delle relative misure previste dal piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu a cura del Commissario straordinario, sono destinati un milione di euro per l'anno 2024, tre milioni di euro per l'anno 2025 e sei milioni di euro per l'anno 2026. Ricordo poi che con il decreto-legge agricoltura n. 63 del 2024 sono state destinate ulteriori risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, per sostenere interventi di supporto e per lo sviluppo della filiera ittica, nonché di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu. con tale previsione è stato predisposto un decreto ministeriale che destina 12 milioni di euro a favore dei consorzi, delle cooperative, delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, nonché delle imprese della pesca lagunare professionale delle acque interne per il rimborso delle spese sostenute per la semina, il ripopolamento e la protezione degli allevamenti. Il testo del citato decreto ha ottenuto l'intesa della Conferenza Stato-Regioni lo scorso 12 settembre ed è in fase di perfezionamento con la relativa sottoscrizione. Inoltre, considerato che i fondi a disposizione non permettono di liquidare il 100 per cento del contributo richiesto dalle suddette imprese, sono stati stanziati ulteriori 15 milioni di euro del cosiddetto Fondo filiere predisposto il relativo decreto ministeriale. Anche tale decreto, ottenuta l'intesa della Conferenza Stato-Regioni il 12 settembre scorso, è in fase di perfezionamento. Occorre tuttavia tener presente che le misure finora stanziate riguardano l'impegno italiano a sostegno del comparto. Pertanto in Europa, durante la riunione dell'ultimo Agrifish abbiamo ribadito l'importanza di strategie comuni, perché le specie invasive e le malattie non rispettano i confini nazionali e richiedono una risposta unitaria. Riguardo poi agli enti e alle istituzioni coinvolte per i quali l'interrogante fa specifica richiesta, segnalo che - come previsto al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 63 del 2024 - il Commissario si può avvalere del supporto tecnico dell'ISPRA, del CNR e del CREA. Da ultimo, informo l'interrogante che il Ministero sta valutando di intraprendere, a valere sul FEAMPA 2021-2027, eventuali azioni per il finanziamento di progetti di studio della biologia della specie, finalizzate non solo al contrasto del crostaceo, crostaceo, ma anche alla creazione di una filiera del granchio blu per il suo utilizzo alimentare come integratori e mangimi per acquacultura e per la commercializzazione e promozione nei confronti del consumatore. Signor Presidente, ringrazio innanzitutto il Sottosegretario e quindi il Governo per la risposta che ci ha voluto dare. Visto che il tema non solo riguarda lo stesso territorio,

dell'acqua si modificano a seguito dei cambiamenti climatici. Questo richiede che le istituzioni, insieme alla scienza, alla ricerca e agli enti che governano i territori, siano in grado tempestivamente di adottare misure di adattamento e di mitigazione.

tutto un comparto ittico che, soprattutto nei comuni di Goro e di Comacchio, determina non solo l'economia, ma anche la tenuta sociale di quel territorio.

alle imprese danneggiate. La stima parla di 40 milioni di euro di danni. Lei ha citato diversi fondi che in qualche modo possono arrivare, ma le imprese e i lavoratori hanno bisogno di risposte immediate. Il Commissario ha bisogno di adottare un piano che risponda oggi e non domani ai danni che vengono subiti dalle imprese e dalle famiglie del territorio. Quello che noi chiediamo al Governo, al di là del decreto e non abbiamo alcun dubbio che il commissario, essendo stato prefetto di quei territori, li conosca bene, agisca con tempestività, dia risposte concrete a quelli che sono i bisogni della popolazione locale, degli imprenditori e di tutto il comparto ittico. a questo tema una strategia europea. Lei ha giustamente citato il fatto che questo tema è stato portato dal Ministro nelle sedi opportune, che sono quelle dell'Unione europea. l'accesso al Fondo europeo FEAMP sia una delle cose da porre sul tavolo. O noi affrontiamo questi temi anche nell'ottica della prevenzione nel contesto europeo o è evidente che saremo sempre costretti a rincorrere la dittatura dell'emergenza.

il comparto ittico e agricolo di quel territorio ha bisogno non di proclami e di annunci, ma di fatti concreti.

Signor Presidente, con gli atti di sindacato ispettivo in oggetto si chiede di conoscere le iniziative che saranno assunte per fare chiarezza in merito all'episodio relativo al rinvenimento, nel fascicolo del dibattimento, prima ancora che il pubblico la sua requisitoria e i difensori argomentassero le loro difese, del dispositivo privo di sottoscrizione recante l'indicazione, oltre che del nominativo dell'imputato e della data della della precedente udienza, anche della decisione di condanna e della pena da irrogare. Sulla base della relazione trasmessa dal presidente della corte d'appello di Firenze, il processo in questione veniva per discussione già alla precedente udienza, ma subiva un rinvio in ragione della presentazione, da parte del difensore dell'imputato, di un'istanza per l'accesso alla giustizia riparativa, sulla quale il collegio si era riservato ogni decisione. All'udienza di rinvio, durante una pausa e nell'assenza dei componenti del collegio e del cancelliere, il difensore dell'imputato, con il consenso del pubblico ministero, esaminava il fascicolo processuale, rinvenendovi il dispositivo completo di alcuni dati, ma non ancora firmato. Ciò induceva il difensore a chiedere un rinvio per poter depositare un'istanza di ricusazione nei confronti del collegio giudicante, istanza poi superata dalla decisione dello stesso collegio di depositare un'istanza di autorizzazione all'astensione, puntualmente concessa. Ciò posto, anche a fronte del clamore mediatico che ha accompagnato la vicenda, lo stesso presidente del tribunale di Firenze, dopo aver autorizzato la richiesta di astensione del collegio della seconda sezione penale, ha ritenuto opportuno portare l'accaduto all'attenzione della procura generale della Corte di cassazione, pur evidenziando come - a suo avviso - non fossero ravvisabili comportamenti scorretti integranti illeciti disciplinari. Sul versante disciplinare, tuttavia, rappresento che la vicenda è all'attenzione delle competenti articolazioni, che valuteranno - come sempre, con la dovuta ponderazione se l'accaduto possa rappresentare o meno un'anomalia del processo e nel processo decisionale idonea a determinare un'effettiva compromissione del diritto di difesa.

salomonica, burocratica e anche evasiva. Se abbiamo dei dubbi che questo sia un illecito disciplinare, allora non so quale possa essere un illecito disciplinare. È del tutto evidente che qualcuno ha scritto la sentenza prima ancora di ascoltare la requisitoria del pubblico ministero e la difesa. Magari si tratterà di un errore. Sappiamo qual è la formula che in situazioni del genere si tende ad accreditare da parte del magistrato incolpato: era solo una minuta preparata dall'ufficio del processo, ma è inaccettabile. Vale il principio che abbiamo declamato tante volte: la giustizia non solo deve essere imparziale, ma deve anche apparire imparziale. La invito caldamente a risollecitare gli uffici del Ministero. il Ministro ha anche la possibilità di attivare l'azione disciplinare. Credo che in casi così eclatanti non si possa far finta di niente, ma si debbano invece adottare delle misure che sono previste dalla legge e non sono eccessivamente punitive. Sappiamo

lapalissiana evidenza e credo che dal Ministero ci si debba attendere delle iniziative più articolate e severe rispetto a quelle illustrate nella sua risposta.

che condividere le preoccupazioni espresse dal collega Zanettin. In un momento storico in cui l'azione requirente - come già dimostrato dalla vicenda Palamara - appare fortemente soggetta ad azioni di condizionamento di raggruppamenti di interesse, è quanto mai opportuno che almeno la figura del giudice mantenga quella terzietà e quella capacità di discernimento giuridico indispensabili a garantire, con la propria autonomia, la pura applicazione della legge alle pendenze processuali. La vicenda fiorentina, del resto, emerge solo grazie a una puntuale e ferma reazione della camera penale di Firenze, che ci ha permesso di esaminare un caso emblematico che risale allo scorso 15 febbraio. Un legale che era in attesa del processo davanti al tribunale scopre, dopo un'attività

Come è noto, il dibattimento si chiude, al termine della discussione, con la dichiarazione di chiusura che fa il Presidente, ai sensi del codice di procedura penale. Quindi, non possiamo permetterci di originare alcun dubbio circa la capacità di amministrare la giustizia. L'episodio denota una visione del processo penale in cui, a volte, le ragioni della difesa vengono intese alla stregua di un inutile orpello cui si possa tranquillamente rinunciare o di cui fare a meno, con conseguenze anche abbastanza delicate, ad esempio per il ruolo e la funzione del difensore. È pertanto opportuno non restare indifferenti alla reiterazione di simili condotte che possono incidere significativamente sul diritto degli imputati e sul giusto processo, con un'intollerabile compromissione della dignità della funzione difensiva e di chi indossa la toga. Bene ha fatto il presidente del tribunale, dottoressa Marilena Rizzo, ad autorizzare quest'attività di accertamento per capire in cosa consisteva quello scritto, se in un'idea di uno dei tre magistrati o magari di un tirocinante, ma di certo non poteva corrispondere a quello che il collegio avrebbe poi dovuto emettere con una sentenza, perché quella è una cosa ben diversa anche dal punto di vista rituale. Noi ci pregiamo di aver sollecitato, attraverso questo intervento ispettivo, la la sua attenzione e quella del Dicastero che lei rappresenta, perché vogliamo che episodi del genere non passino assolutamente inosservati e siano invece un po' di spunto per il comportamento e la condotta che spesso richiediamo ai nuovi giovani magistrati che, in maniera integerrima, è opportuno che colmino delle lacune anche di loro predecessori che non hanno dimostrato quella integerrima condotta che anche il Presidente della Repubblica più volte ha ricordato essere indispensabile nell'esercizio della funzione giudiziaria.

senatori, con riguardo alle criticità segnalate dal tribunale di sorveglianza di Roma, ricordo che per il Ministero della giustizia - come ribadito in varie occasioni - costituisce un obiettivo primario assicurare una giustizia efficace ed efficiente attraverso anche politiche di valorizzazione delle risorse umane. In quest'ottica, dunque, mi accingo ad illustrare le iniziative assunte per far fronte alle lamentate criticità, sia per quanto riguarda il personale amministrativo che l'organico della magistratura. Relativamente alla situazione del tribunale di sorveglianza di Roma, si registra una scopertura del 31 per cento, ove, a fronte di una dotazione organica di 78 unità, prestano servizio 54 risorse. Il dato, tuttavia, non tiene conto dell'assenza per distacco di altro ufficio di due assistenti giudiziari e di un direttore e di un altro distacco di ufficio di un assistente giudiziario. Le vacanze registrate nei vari profili interessano le seguenti figure professionali: assistente giudiziario, 5 vacanze su 20 in organico; cancelliere, 12 vacanze su 14 in organico; direttore, 1 vacanza su 6 posti; conducente di automezzi, 7 vacanze su 9 posti. Le figure dell'assistente alla vigilanza dei locali e al servizio automezzi e dell'ausiliario del contabile risultano coperte. Di contro, si evidenzia la presenza di posizioni in sovrannumero:

Passando alle attività assunzionali realizzate per il tribunale di sorveglianza di Roma nell'arco temporale riferibile a questo Governo, 2022-2024, si segnala che sono state effettuate 8 assunzioni ordinarie, 3 stabilizzazioni di operatori giudiziari, 2 riqualificazioni di ausiliari in operatori giudiziari, 6 riqualificazioni cancellieri in funzionari giudiziari. Inoltre, per il distretto di Roma è di prossima pubblicazione un bando di concorso per 1.000 posti per il profilo di conducente di automezzi e, quindi, area assistenti. È stato disposto, con avviso del 31 maggio, lo scorrimento degli idonei del concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale di area assistenti. La procedura è *in itinere* per il distretto di Roma sono riservati 278 posti nel profilo amministrativo, di cui 226 nel solo circondario di Roma. È in programma la pubblicazione di un corso concorso SNA (Scuola nazionale dell'amministrazione) per l'assunzione di ulteriori 70 unità di dirigenti di seconda fascia. Per fronteggiare le ulteriori criticità che nel frattempo dovessero sopravvenire - con tale espressione mi riferisco al pensionamento del personale, ovvero alle altre situazioni di carattere temporaneo, come maternità, malattia, eccetera - l'organico dell'ufficio interessato potrà essere implementato facendo ricorso all'istituto della mobilità temporanea del personale, previsto dall'accordo sulla mobilità interna del personale. Per il futuro, infine, si segnala la disponibilità del Ministero a procedere alla sottoscrizione di accordi quadro con le Regioni interessate, aventi ad oggetto anche forme di collaborazione in tema di selezione e reclutamento di personale con procedure concorsuali uniche per far fronte ai reciproci e coincidenti fabbisogni. Le tematiche relative alla copertura delle piante organiche del personale di magistratura sono invece un'attribuzione - come sapete - del Consiglio superiore della magistratura, a cui spetta assumere le relative determinazioni. Tuttavia, relativamente ai profili di competenza di questo Ministero della giustizia, si evidenzia che la riforma della geografia giudiziaria ha determinato rilevanti modifiche all'assetto dei tribunali di sorveglianza, considerato considerato che la competenza territoriale di tali uffici si estende alle circoscrizioni di due o più tribunali. In tale contesto, sono stati realizzati nell'arco temporale 2014-2016 settoriali e mirati interventi di adeguamento delle relative piante: si fa riferimento ai decreti ministeriali del 2014, 2015 e 2016, che hanno determinato un aumento di complessive 31 unità di personale di magistratura. Si rimarca il deciso rafforzamento dell'organico della magistratura di sorveglianza avvenuto mediante l'impegno profuso da questo Governo, che ha portato all'attribuzione di 21 unità con il decreto ministeriale 23 novembre 2022. Anche di recente, in un'ottica di leale collaborazione, il Ministro della giustizia ha rappresentato al Consiglio superiore della magistratura di mettere a concorso i posti sopra individuati al fine di assicurare una copertura completa dell'organico. In definitiva, gli uffici di sorveglianza hanno beneficiato, nell'ultimo decennio, di un deciso rafforzamento dei relativi organici: specificatamente, l'aumento del personale di magistratura è stato di complessive 73 unità, di cui 42 per effetto dei recenti e ravvicinati interventi ministeriali, l'ultimo dei quali realizzato nel mese di novembre 2022. Si tratta quindi di un incremento del 36 per cento rispetto alla pianta organica preesistente, che non ha eguali in altre tipologie di ufficio. L'opera di rafforzamento ha riguardato anche gli uffici di sorveglianza del distretto di Roma. Il citato decreto ministeriale 14 settembre 2020 ha previsto, tra l'altro, l'aumento di una unità per l'ufficio di sorveglianza di Roma. L'intero distretto aveva già beneficiato in tempi recenti di due unità complessive per effetto dei decreti ministeriali del 2014 e del 2015, specificatamente assegnati in ragione di una unità ciascuna agli uffici di sorveglianza di Viterbo e Frosinone. Da ultimo, con decreto ministeriale 23 novembre 2022 è stata disposta un'ulteriore attribuzione di due unità all'ufficio di sorveglianza di Roma, con un incremento complessivo del 20 per cento della pianta organica nel periodo di riferimento.

in una incapacità e anche in una mancanza di volontà del Governo e del Ministero che questa mattina lo rappresenta qui in Aula di voler affrontare seriamente la questione delle carceri e, nel caso specifico, la questione collegata della magistratura di sorveglianza. Noi siamo partiti mesi fa, nel presentare questa interrogazione,

Questo grido d'allarme sulla drammatica situazione dello stato della magistratura di sorveglianza venne raccolto dalla presidente del del tribunale di sorveglianza di Roma, la dottoressa Marina Finiti, la quale mandò una risposta chiedendo a sua volta, quasi supplicando il Governo, il CSM e tutti i soggetti preposti,

avremmo potuto presentarla per tanti altri tribunali di sorveglianza del nostro Paese. Le vostre risposte a questa situazione sono state intanto tutte declinate al futuro (faremo, abbiamo in programma, vedremo), quando invece

decreto carceri, che è un po' - come ha detto Antigone - come provare a ridipingere le pareti di una casa quando essa sta crollando dalle fondamenta. E mi riferisco al al sistema carcerario italiano: suicidi, sovraffollamento, tutte cose di cui abbiamo parlato anche in quest'Aula. Avete aggravato la situazione anche della magistratura di sorveglianza nella relazione con i detenuti, in un momento di fortissima tensione negli istituti di pena. Lo diceva molto bene il magistrato di sorveglianza Gianfilippi in una delle audizioni che abbiamo svolto, ma lo diceva anche il coordinamento dei magistrati di sorveglianza, che ha presentato un documento

semestrali, che i magistrati di sorveglianza elaboravano per valutare l'andamento del trattamento, valutando cioè la qualità e la quantità del percorso di recupero che ogni detenuto aveva deciso di intraprendere in quelle situazioni. Per un detenuto questo è fondamentale: è come una pagella quadrimestrale in una scuola. Voi avete abolito le pagelle quadrimestrali; avete assegnato al magistrato di sorveglianza solo il giudizio finale in vista di quando scatterebbe scatterebbe la possibilità della liberazione anticipata, creando un'ulteriore tensione. Quella pagella, quel giudizio temporale serviva - e serve - anche al detenuto a capire se il suo percorso è tale da poter poi meritare quell'auspicata e agognata liberazione anticipata. L'avete abolita. I magistrati di sorveglianza hanno protestato, ma anche questa protesta sacrosanta è andata nella vostra indifferenza. Signora Presidente,

in una situazione del genere, quando nominerete il nuovo Garante, con quali criteri, ne parlerete col Parlamento, cosa che non avete fatto l'altra volta? Darete un segnale di serietà anche su questo punto che, con la vostra politica carceraria, non state dando? *(Applausi)*.

una nuova finestra"). Comunico che il Parlamento in seduta comune è convocato martedì 24 settembre 2024, alle ore 12,30, con all'ordine del giorno la votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

*(IV-C-RE)*. Signor Ministro, c'è una realtà dei fatti e c'è la propaganda del Governo. La propaganda del Governo è che questo è un Paese da due anni più sicuro. La realtà dei fatti, purtroppo, dice il contrario e lo diciamo con dispiacere. I dati dicono che, da quando c'è il Governo Meloni, ci sono più reati e c'è meno sicurezza. Uno potrebbe pensare che questo derivi dall'aumento delle previsioni normative, perché è noto che in una iperproduzione legislativa, da quello di *rave party* in poi, vi siete inventati i reati più strani. Ma in realtà i numeri che ci vengono offerti

(non di *rave party*) e che aumentano persino gli omicidi volontari rispetto al 2022 e rispetto al 2019. Signor Ministro, nell'augurarle buon lavoro e nel dirle che sui temi della pubblica sicurezza ovviamente siamo dalla sua parte, le diciamo anche che quest'estate siamo rimasti colpiti: una volta la Presidente del Consiglio evocava un complotto, una volta il Ministro - lei stesso - parlava di trappolone - penso che scopriremo, prima o poi, che il trappolone e il complotto ve li siete fatti da soli - ma il concetto di fondo è che, mentre il Palazzo discute di complotti e trappoloni, la sicurezza del ceto medio, degli ultimi o forse dei penultimi, è messa in discussione. Da quando ci siete voi, ci sono più reati. Che cosa intendete fare per cambiare linea?

alla sicurezza nelle città, attivando un *forum* con i sindaci delle Città metropolitane sui temi della sicurezza urbana e presiedendo personalmente comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica in molti Capoluoghi. I dati, in realtà, indicano che nel primo semestre 2024 i delitti sono calati sul territorio nazionale complessivamente dell'1,1 per cento rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, con una rilevante flessione, tra l'altro, proprio degli omicidi volontari, diminuiti del 28 Nello stesso periodo sono stati oltre 400.000 i soggetti denunziati ed arrestati, di cui circa 139.000 stranieri. Vista l'incidenza dei reati commessi da migranti irregolari, un forte impulso è stato dato proprio all'attività di rimpatrio degli stessi, anche grazie ad operazioni straordinarie realizzate dalle questure. Sono 3.724 i rimpatri effettuati dall'inizio dell'anno ad oggi, a fronte dei 3.164 dello stesso periodo dello scorso anno. Confidiamo in un progressivo ulteriore incremento di questi dati in relazione alla prossima riattivazione di alcune centinaia di posti nei centri per il rimpatrio, danneggiati dagli stessi occupanti. I risultati ottenuti sono frutto della sempre più incisiva attività di presidio e controllo del territorio assicurata dalle Forze di polizia, che ha portato a un aumento delle persone controllate del 14,7 per cento rispetto all'anno precedente. *trend* è confermato in crescita nei primi sei mesi di quest'anno, con un incremento del 3,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023. Nelle grandi città la realizzazione sistematica di operazioni interforze, che noi abbiamo definito ad alto impatto, sta inoltre restituendo risultati molto positivi in termini di capacità di controllo del territorio, di prevenzione e di contrasto di ogni forma di illegalità. A partire dal gennaio 2023 ne sono state realizzate oltre 2.000, con l'impiego di 91.000 unità delle Forze di polizia; sono state controllate 750.000 persone, di cui 263.000 stranieri, 1.400 i soggetti arrestati e oltre 9.000 denunziati. Si tratta di iniziative che si inseriscono nel contesto di un più ampio disegno finalizzato a potenziare la presenza delle Forze dell'ordine nei luoghi pubblici ad elevata concentrazione di persone. Con l'ultima legge di bilancio abbiamo infatti rafforzato la presenza dei militari nelle stazioni ferroviarie, finanziando un'aliquota di personale dedicato di 800 unità e abbiamo incrementato il contingente dei militari dell'operazione Strade sicure, portando a 6.000 le unità rispetto alle 5.000 originariamente previste. L'obiettivo è quello di rendere ancora più incisiva l'azione di presidio e controllo delle nostre città grazie al Fondo per le assunzioni, previsto nella legge di bilancio per l'anno 2023, e agli stanziamenti assicurati ancora per gli anni a venire. Stiamo attuando un'inversione di tendenza storica rispetto ai tagli operati nel passato da Governi precedenti, aumentando la presenza delle Forze dell'ordine nelle nostre città e ringiovanendo gli organici. mia intenzione, pertanto, continuare ad assicurare il necessario sostegno alle Forze di polizia con ulteriori risorse, che auspico possano essere individuate nella prossima legge di bilancio, e a proseguire con politiche di sicurezza ad ampio raggio anche grazie

Ella si è prodotto in una serie di dati e numeri che non colgono il punto di vista molto chiaro che l'ufficio del Viminale ha espresso alla pubblica opinione. Dal 2013 tutti gli anni i reati sono diminuiti. E ripeto: tutti gli anni dal 2013 fino al 2022. Nel 2023 hanno ricominciato a crescere. Sono veri questi dati o dobbiamo dubitare del Viminale? Io non dubito del Viminale. Io ho fiducia nelle Forze dell'ordine e nella Polizia, in quelli che stanno sul territorio e in quelli che stanno negli uffici del Palazzo, al piano dell'ascensore o da un'altra parte. Io ho fiducia nella Polizia. Forse il fatto che lei non dica la verità, e cioè che in questi due anni qualcosa è andato male, è comprensibile dal punto di vista politico. Ma lei è un servitore dello Stato. Ha fatto riferimento al taglio dei Governi precedenti. Lei era al Viminale quando il nostro Governo ha riaperto contro il blocco delle assunzioni e contro il blocco degli stipendi. Signor Ministro, la sicurezza non è né di destra né di sinistra: è di tutti, degli ultimi e dei penultimi, delle ragazze che in stazione non ce la fanno *(Applausi)*, dei cittadini che prendono la metropolitana perché non hanno i soldi per il taxi, è di quelli di cui voi volete il voto e a cui poi voi raccontate - come ha fatto lei oggi una sfilza di numeri privi di significato. Siccome io ho stima nei suoi confronti, signor Ministro, la prego: la prossima volta anziché parlare di altro, risponda nel merito e, se mi posso permettere, non ci racconti la storia dei trappoloni e dei complotti. Occupatevi dei problemi degli italiani, non dei fantasmi dei vostri Ministri.

Signor Presidente, Governo, Ministro, colleghi, come è noto, il 14 settembre scorso il pubblico ministero di Palermo, nell'ambito del processo Open Arms, ha chiesto una condanna a sei anni di reclusione per l'allora - è ancora Ministro, ma in un altro Dicastero - ministro Salvini. Non ritorno sul merito della richiesta e della faccenda, di cui si è ampiamente dibattuto. L'interrogazione di oggi volge lo sguardo su due effetti collaterali di questa richiesta. In particolare, mi riferisco alla dichiarazione di solidarietà che tanti membri del Governo - quasi tutti - hanno fatto al ministro Salvini. Però nello specifico, Ministro, abbiamo visto una sua dichiarazione in cui, oltre a esprimere solidarietà a una persona sotto processo - questo mi sembra sia del tutto lecito - ribadisce, con una frase molto precisa, il rischio che una condanna a sei anni di carcere per aver fatto fino in fondo il proprio dovere nel contrasto all'immigrazione irregolare sia un'evidente e macroscopica stortura e un'ingiustizia per lui e per il suo Paese. Io personalmente ritengo - ma ovviamente chiedo a lei la sua opinione - che un Ministro della Repubblica, essendo Ministro della Repubblica e quindi di tutti noi, possa esprimere un moto di solidarietà verso un collega che ha una situazione complicata, ma dovrebbe cercare in qualche modo di limitare l'acuirsi di uno scontro fra poteri dello Stato. Ritengo che, da Ministro della Repubblica, si debba cercare di evitare di alimentare una visione per cui il potere esecutivo si contrappone Il ministro Salvini avrà un processo, con tutte le garanzie del giusto processo, e sarà la magistratura a determinare se, anche nell'eventualità di un'attività esclusivamente doverosa di contrasto all'immigrazione, sia stato commesso un reato. Ancor più deprecabile - mi permetto di dire - è il fatto che quella sua dichiarazione sia stata postata sui canali *social* non suoi, nella sua funzione di Ministro, ma del Viminale, perché ritengo che un Ministero che ha dei suoi canali di comunicazione debba utilizzarli per evidenziare l'attività, anche politica, del Ministero e del Ministro, ma non certamente per fare politica. di riferirmi a casi di personalità di precedenti Governi, anche appartenenti al Gruppo politico interrogante, che durante l'incarico ministeriale hanno rilanciato sul *web*, tramite canali istituzionali, proprie opinioni politiche, anche poco attinenti al mandato ricoperto. Attribuisco piuttosto il significato di questa interrogazione al tentativo, che ricorre più volte, di rinunziare a contraddire il Governo nel merito delle questioni affrontate, probabilmente per scarsità di argomenti convincenti, preferendo cercare ragioni per contestarne la legittimazione a esprimere le proprie posizioni. Nel caso di specie, innanzitutto preciso che non ho mai assolutamente detto che sia ingiusta l'attività della magistratura. Prego di controllare bene il testo e il significato della mia dichiarazione. La magistratura requirente e giudicante fa anche in questo caso il proprio lavoro, secondo quanto gli è stato istituzionalmente consegnato. Infatti - come anche molti opinionisti indipendenti hanno sottolineato è stato ingiusto, per quanto legittimo, consegnare alla giurisdizione penale l'attività istituzionale di un Ministro, volta al contenimento dell'immigrazione irregolare, da parte di Gruppi politici parlamentari che, in altri analoghi precedenti casi, non solo si erano espressi in senso diametralmente opposto, ma avevano anche rivendicato il valore politico e la riconducibilità ad azioni di Governo delle medesime iniziative da parte dello stesso Ministro, in alcuni casi intestandosi persino il reale merito di tali iniziative. Peraltro a tale situazione, dal significato del messaggio che ne derivò, fece seguito un'immediata ripresa dei numeri crescenti di arrivi di migranti irregolari sulle nostre coste, che solo con l'impegno dell'attuale Esecutivo, dopo alcuni anni, si sta contrastando con efficacia e con risultati che sono sotto gli occhi di tutti: ad oggi meno 65 per cento di ingressi irregolari rispetto all'anno scorso, ma anche meno 34 per cento rispetto al 2022. È questo - io ritengo - l'interesse esclusivamente istituzionale che da attuale Ministro dell'interno annetto all'intera vicenda. E non mancheremo alcuna occasione per ribadire ai trafficanti di esseri umani che il Governo Meloni continuerà in ogni direzione a contrastare il loro vergognoso mercato criminale, assecondando da parte nostra, per converso, corridoi di ingressi legali per motivi umanitari e di lavoro, anche in questo caso con numeri mai registrati nel recente passato. Signor Presidente, penso che diciannove mesi di fila di calo della produzione industriale; i dati sull'occupazione che sembrano così buoni, ma in realtà denotano un calo delle ore lavorate e quindi una diminuzione dei lavoratori; i salari che vedono il nostro Paese al penultimo posto in Europa per la loro crescita e la fallimentare politica europea di questo Governo sono questioni che ogni giorno rilanciamo, perché di argomenti per contrastare politicamente e nei fatti questo Governo Ve ne sono anche altri, come quelli illustrati nella mia interrogazione. Penso che, rispetto all'opinione che si ha sul processo di Salvini, ci sia la massima libertà ed io ho rispetto di tutte le opinioni. Avrei preferito sentire un «sì, scusate» sul sito del Ministero dell'interno e un «forse era meglio che non vi fosse una mia dichiarazione politica», a prescindere da chi l'ha fatto prima e da chi lo farà dopo, perché ciascuno poi è responsabile delle proprie cose. Quindi, il Ministro ha perso l'occasione per ammettere semplicemente che forse è stato un errore e che cercherà di stare più attento nella comunicazione del Ministero. Su tutto il resto, come sulla lotta all'immigrazione, possiamo confrontarci, ma la domanda era puntuale e specifica. Un po' come nella risposta precedente, lei ha cercato in qualche modo di dribblarla. Ripeto: chiedere scusa in questo Paese credo sia una pratica poco frequentata,

Signor Presidente, ministro Piantedosi, da emiliana e siccome il quesito riguarda l'Emilia-Romagna, permettetemi di cogliere l'occasione - mi sembra doveroso - per rivolgere la mia vicinanza, e penso anche quella dell'Assemblea e vostra, alla popolazione dell'Emilia-Romagna colpita dall'alluvione di questa notte. Ringrazio tutti i soccorritori, i volontari e le Forze dell'ordine che stanno naturalmente lavorando per soccorrere la popolazione. Veniamo al quesito. Ho voluto presentare questa interrogazione perché purtroppo la situazione delle città, dei cittadini e delle attività commerciali dell'Emilia-Romagna è ogni giorno preoccupante per quanto riguarda la sicurezza. La città e le piazze emiliane, che di solito sono un luogo di socialità e spesso di attività culturali, sono state trasformate, specialmente di notte, in luoghi di delinquenza e violenza. I capoluoghi di Provincia, anche i piccoli Comuni e le piccole città del territorio, sono oggetto di furti, rapine e risse, con interi quartieri in mano alla microcriminalità, in cui si percepisce un livello di insicurezza altissimo. La diffusione incontrollata di spaccio di droga ha raggiunto livelli allarmanti. È un fenomeno criminale che si svolge in pieno giorno nelle vie adiacenti alle stazioni ferroviarie, ma anche in zone frequentate da famiglie e da ragazzi, addirittura davanti alle scuole. Dal 2014, le amministrazioni comunali di diverse città in Emilia-Romagna hanno inaugurato campagne di accoglienza che, nel tempo, hanno portato però a risultati fortemente negativi e l'aumento tangibile della criminalità. La stessa cosa per quanto riguarda l'accoglienza di minori stranieri, che trovano immediata accoglienza, ma poi vengono lasciati soli e abbracciano direttamente la criminalità, facendo parte anche di baby-gang. Ci sono vere e proprie organizzazioni che gestiscono il *racket* dei posti letto degli immigrati irregolari e nei centri di accoglienza straordinaria succede

Presidente, anch'io colgo l'occasione per rivolgere a nome mio e del Governo un pensiero di vicinanza e di solidarietà alla popolazione dell'Emilia-Romagna, che in queste ore sta fronteggiando una nuova grave alluvione. In Emilia-Romagna, come nel resto del Paese, le prefetture sono costantemente impegnate a coordinare l'azione di prevenzione e contrasto poste in essere dalle Forze di polizia sulla base delle specifiche esigenze territoriali e con metodologie di intervento in grado di valorizzare le esperienze informative e investigative. Tra le città capoluogo dove mi sono recato per presiedere personalmente i comitati provinciali non poteva non esserci Bologna, peraltro città alla quale sono profondamente legato per ragioni professionali e di vita. Altri momenti di confronto e di approfondimento sono stati da me voluti anche a Modena e Ravenna. A Bologna, dove sono stato in più occasioni, è stato anche sottoscritto il nuovo patto per la sicurezza urbana integrato: un accordo di durata biennale tra prefettura e Comune capoluogo che delinea una cornice organica di misure finalizzate a fornire risposte mirate in settori di intervento ritenuti prioritari per la sicurezza e per contrastare situazioni di degrado o di illegalità, in linea con le direttive da me impartite per incrementare i servizi di presidio e di controllo del territorio. Le Forze di polizia, anche in questa Regione, sono state costantemente impegnate in un'attività che ha portato all'intensificazione dei controlli sulle persone, sui veicoli, sugli esercizi commerciali e ricettivi; al sequestro di stupefacenti, di merce insicura, contraffatta o provento di reato; all'adozione di provvedimenti di espulsione a carico di stranieri irregolari e di misure di prevenzione personale. In questo impegno, dall'inizio dell'anno ad oggi, sono stati messi a disposizione dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza di quella Regione oltre 3.300 equipaggi dei reparti prevenzione crimine della Polizia di Stato, con l'impiego aggiuntivo di più di 10.000 unità di personale, oltre alle forze territoriali. Nelle città di Bologna e Modena vengono inoltre sistematicamente effettuate operazioni cosiddette ad alto impatto: per l'anno in corso nelle due città sono stati già realizzati quarantaquattro servizi con tali modalità, con uno specifico *focus* su stazioni ferroviarie e aree limitrofe, con importanti risultati in termini di persone identificate e arrestate. Si tratta di una strategia di intervento articolata sul piano operativo e alla quale stiamo assicurando la necessaria continuità in termini di uomini e mezzi, anche con l'incremento dei militari di Strade sicure, che vede oggi impegnate 226 unità. Siamo convinti che tale azione possa essere ulteriormente rafforzata, sicuramente grazie ai nuovi strumenti normativi contenuti nel disegno di legge per la sicurezza pubblica approvato ieri alla Camera dei deputati. Ricordo che le nuove misure consentiranno di contrastare più efficacemente alcune forme di criminalità che interessano proprio le aree urbane e che incidono sulla percezione di sicurezza, come le occupazioni abusive di immobili, le truffe, i borseggi e i reati commessi in luoghi ad alta densità di persone. Con questo provvedimento rafforziamo la tutela anche degli operatori delle Forze di polizia, che devono poter lavorare con serenità. Tra le nuove misure introdotte dall'esame alla Camera voglio segnalare peraltro il miglioramento degli strumenti di assistenza legale a favore di chi viene indagato per fatti avvenuti in servizio e le *bodycam* a garanzia di coloro che sono impegnati in servizio di ordine pubblico e di controllo del territorio.

prevenire la loro tutela. Ecco perché quanto approvato con il decreto sicurezza alla Camera è rilevante anche dal punto di vista della sicurezza degli operatori. Mi riferisco, ad esempio, alle *bodycam*; alla copertura delle spese legali fino a 10.000 euro per ogni grado di giudizio nel caso siano imputati o indagati; alle pene più severe per chi usa violenza o minaccia a un ufficiale o

l'ordine laddove si è radicata la criminalità, ed è quello che stiamo facendo e che state facendo come Governo. Naturalmente deve essere innalzato anche il livello di sicurezza percepito e, quindi, è importante anche la comunicazione ai cittadini.

*(PD-IDP)*. Signor Ministro, una persona in piazza minaccia e mette le mani addosso a un giornalista dopo averne insultati pubblicamente altri. Nella stessa piazza quella stessa persona lancia sputi a un cittadino. La medesima persona poi minaccia in un'aula consiliare dirigenti e dipendenti comunali; insulta e intimidisce consiglieri comunali con aggressività, costringendo i vigili urbani a cinturarlo e a bloccarlo. Pronuncia ripetutamente in quell'aula frasi e insulti sessisti. Lei dirà che questa persona minaccia l'ordine pubblico, che bisogna prevenire e contrastare questi comportamenti. Il problema è che questi gesti da energumeno appartengono a un pubblico ufficiale: il sindaco di Terni. Hanno messo a rischio la coesione sociale in quella città, la convivenza civile e la stessa agibilità democratica in una città di forti tradizioni democratiche e civili, come Terni, e l'agibilità dello stesso consiglio comunale, organo eletto dal popolo, i cui membri devono essere garantiti nell'esercizio del mandato. Questo sindaco, che si chiama Stefano Bandecchi, ha violato ogni regola democratica, mettendo in crisi l'organo, costringendo alcuni consiglieri comunali a presentare perfino denunce per minacce e intimidazioni ricevute, mozioni all'unanimità di censura, di condanna da parte del consiglio regionale dell'Umbria; la

il mio intervento dicendo che da quando abbiamo presentato l'interrogazione sono accaduti dei fatti nuovi, per esempio c'è stata la chiusura delle indagini per un'inchiesta molto seria, della Guardia di finanza e della procura di Roma, che aveva provocato perfino il sequestro cautelativo di 22 milioni di euro a Bandecchi per evasione fiscale e per violazione delle norme delle università private. C'è un tema di conflitto di interessi legato al nuovo stadio e a una clinica privata che lui vorrebbe costruire; si è dovuto dimettere da presidente della Ternana, sta cercando di vendere la società a chissà quali soggetti poco affidabili, ma c'è un grande tema di incompatibilità e di conflitto d'interesse. davvero una presenza inquinante della democrazia. Mi dispiace che la destra, che lo ha combattuto in questo anno, nei giorni scorsi abbia stretto un accordo politico per le elezioni regionali con questo personaggio e il suo movimento. Non è questo, ovviamente, che voglio imputare a lei, ma a lei chiediamo risposte sulla garanzia garanzia dell'agibilità democratica in quella città e in quel consiglio comunale. Signor Presidente, prima di tutto preciso immediatamente che, rispetto all'alterco avvenuto il 5 settembre scorso nei pressi del palazzo municipale tra il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ed un opinionista sportivo locale, non risultano ad oggi essere state presentate denunce o querele da parte degli interessati. Per quanto attiene ai casi per i quali lo stesso sindaco è stato oggetto di esposti e querele alla competente procura della Repubblica, mi attengo ai reati che possono avere un'incidenza rispetto alle valutazioni che possono essere fatte ai sensi del testo unico degli enti locali; per reati quali violenza, minaccia e oltraggio a un corpo politico, amministrativo, giudiziario si attendono gli esiti degli accertamenti dell'autorità giudiziaria competente, prima dei quali non è possibile fare ogni altra eventuale e consentita valutazione. Assicuro comunque che, come come lei saprà, ogni situazione concernente la possibile sussistenza di cause ostative all'esercizio del mandato amministrativo da parte di amministratori locali è normalmente e puntualmente oggetto di attenzione da parte del Ministero dell'interno, anche per il tramite delle competenti prefetture.

che altro deve accadere. Dei consiglieri comunali sono stati minacciati con violenza, intimiditi, costretti a uscire dall'aula perché non possono rispondere a violenza con la violenza e sono stati costretti a fare delle denunce; sull'agibilità democratica in un organo eletto dal popolo, perché quelle persone, quei consiglieri comunali sono eletti dal popolo e hanno il diritto di svolgere democraticamente il proprio mandato. Ebbene, nell'attesa di tutti gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e anche dell'evoluzione delle querele che sono state state presentate, credo che il prefetto e il Viminale abbiano il dovere di fare anche qualcosa di più, di andare a vedere davvero concretamente quello che sta succedendo in quella città. Infine, signor Presidente, prima ho fatto un accenno a quel

Il candidato sindaco di Fratelli d'Italia Masselli e la dirigente scolastica Fabrizi, entrambi consiglieri di Fratelli d'Italia, hanno lasciato, per protesta e dignità, il loro partito contro questo accordo, che è veramente osceno. Esprimo, per così dire, solidarietà a queste persone che hanno fatto questo gesto, ma al tempo stesso credo che, anche in vista delle regionali, non si possa dare fiducia e fare accordi con chi inquina la convivenza civile e democratica di quella città e anche di quella Regione.

questa iniziativa si svolge all'interno della più ampia iniziativa che Forza Italia ha promosso quest'estate con un comune sentire operativo con il Partito radicale italiano, denominata «Estate in carcere». C'è stata, signor Ministro, una mobilitazione con visite di parlamentari, consiglieri regionali, amministratori e militanti negli istituti di pena, volta a verificare le reali condizioni delle persone private della libertà personale a confrontarsi con i dirigenti, gli operatori, la Polizia penitenziaria, i magistrati di sorveglianza, per redigere *report* dedicati alle singole strutture che, tra l'altro, a a giorni verranno presentati pubblicamente, sempre con intento particolarmente costruttivo e positivo, cercando di dare un contributo che possa servire a migliorare le condizioni della popolazione carceraria. Nell'ambito di questa iniziativa, sono stati visitati anche gli istituti penitenziari di Brescia, che consistono nella casa circondariale Canton Mombello (il vecchio Nerio Fischione, chiamato da noi bresciani Canton Mombello) e la casa di reclusione di Brescia Verziano. Con il collega onorevole Casasco abbiamo visitato entrambe le strutture e parlato a lungo con la direttrice, che vive una situazione chiaramente di grave difficoltà, ma con una strana anomalia: questi due istituti

un vero modello, che, grazie anche agli spazi che ha a disposizione in periferia, ha la possibilità davvero di essere punto di riferimento per nuove iniziative. oggi accade che il Ministero che lei rappresenta ha elaborato l'esigenza di sostituire il carcere di Canton Mombello con un nuovo carcere che si era localizzato a Verziano, ma il MIT - questo vale per la passata legislatura, a cui risale l'iniziativa, che però prosegue - ha avuto la brillante idea di posizionare questa nuova struttura all'interno del campo da calcio della struttura già esistente del sedime di Verziano. Verziano. È evidente che questo porterebbe a creare una anomalia negativa dentro un'esperienza positiva che è quella del Verziano, perché venendo meno gli spazi esterni ci sarebbe un aggravio aggravio del sovraffollamento che abbiamo a Canton Mombello. In più questa iniziativa non chiuderebbe Canton Mombello, non darebbe la possibilità di superare un bubbone che non ha rispetto della tradizione italiana, del nostro comune sentire rispetto alle condizioni carcerarie. Gli interroganti, quindi, chiedono di sapere quale sia in proposito la posizione del Ministro in indirizzo, considerato che a Brescia, realizzando le strutture rappresentate fuori dal sedime, quindi nelle aree adiacenti disponibili, si possono creare le condizioni per garantire la detenzione in ambienti non degradati, necessarie a guidare il reinserimento del detenuto dopo aver scontato la pena, noi ci auguriamo in modo dignitoso.

Il discorso, ovviamente è molto più ampio, essendo nota la situazione di criticità delle nostre strutture penitenziarie. per quanto riguarda l'edilizia, da una situazione che si è sedimentata nei decenni perché non sono stati costruiti nuovi edifici carcerari, né ristrutturati abbastanza quelli vecchi.

circa un quinto di detenuti in attesa di giudizio e circa un altro quinto di detenuti per reati legati alla tossicodipendenza. Da un punto di vista strategico, stiamo lavorando in questi tre settori: per quanto riguarda gli stranieri, cercando, nei limiti del possibile, di far loro scontare la pena nei Paesi di origine; per quanto riguarda i tossicodipendenti, che più che essere criminali sono essenzialmente dei malati, di trovare delle strutture alternative per l'esecuzione della pena, quindi comunità e altro; per quanto riguarda i detenuti in custodia cautelare, rivedendo i criteri della detenzione cosiddetta preventiva. Infine, per quanto riguarda l'edilizia carceraria, che è poi la cosa che ci interessa di più,

che avrà la possibilità di accelerare, sia dal punto di vista burocratico sia dal punto di vista organizzativo, la ristrutturazione di queste carceri, che ripeto, in parte sono anziane, in parte sono fatiscenti e in parte devono essere costruite. Per quanto riguarda nello specifico l'istituto di Brescia di cui lei ha parlato, l'ipotesi progettuale dell'istituto Verziano, sviluppata per l'ampliamento, che contempla allo stato una capacità detentiva pari a 220 posti, consentirà di mantenere adeguati spazi per l'espletamento delle fondamentali attività trattamentali della popolazione detenuta. Faccio presente che il concetto di spazio che lei ha giustamente evocato per noi è fondamentale. Lo spazio infatti nell'ambito del carcere consente quelle due attività, il lavoro e lo sport, che sono deflattive sia dal punto di vista della tensione psicologica sia dal punto di vista dell'attitudine a reiterare i reati. Per quanto riguarda i fondi occorrenti per la realizzazione degli interventi, sebbene l'amministrazione penitenziaria abbia comunicato la disponibilità a poter sostenere a propria cura e spese gli altri due lotti funzionali, il MIT, in sede di riprogrammazione delle risorse finanziarie in materia di edilizia, ha previsto la copertura finanziaria a suo carico dell'intero intervento. La previsione presuntiva di spesa complessiva è di circa 40 milioni e 500.000 euro. Ciò al netto dell'impegno che è già stato assunto dal Governo per un nuovo progetto di edilizia carceraria a Verziano più capiente rispetto a quello attualmente finanziato.

dalle sue buone intenzioni e dalla visione che è assolutamente comune e condivisa. C'è un problema. Noi siamo abituati, purtroppo da tanti anni, al fatto che i progetti partono con una buona intenzione e, quando poi nascono male, vanno avanti perché non si fermano più. In questo caso si tratta di un progetto positivo che va però spostato. Essendo in periferia, le aree adiacenti sono totalmente disponibili. Noi dobbiamo spostare questo progetto dal sedime interno di Verziano all'esterno.

alla costruzione degli spazi solo in termini di metri quadrati. Dobbiamo avere più metri quadrati possibili per poter dare più risposte possibili in termini di cifre, di metri quadrati per detenuto. Non è così che raggiungiamo l'obiettivo, perché in questo caso, se dovessimo consumare il sedime interno di questo carcere e, in più, non si dovesse chiudere Canton Mombello, avremmo il terzo carcere a Brescia che sarebbe un terzo problema. Il primo lo abbiamo già,

Signor Presidente, ringrazio il Ministro per la presenza in Aula. Apprendiamo di recente dalla stampa che due giornalisti, Nello Trocchia e Sara Giudice, si sarebbero resi autori di violenze sessuali ai danni di una giovane collega giornalista, che per tali fatti ha sporto denuncia. Nella denuncia si precisa che le presunte violenze hanno avuto luogo nella notte del 29 gennaio 2023 in un taxi. La denunciante ipotizza anche di essere stata vittima di somministrazione della cosiddetta droga dello stupro. In seguito alla denuncia si aprono le indagini e il pubblico ministero procede, tra l'altro, ad ascoltare più volte i due denunciati, ma, sempre secondo quanto riferito dalla denunciante, omette di ascoltare la parte offesa, in palese violazione della legge n. 69 del 2019, meglio conosciuta come codice rosso, che prevede tassativamente l'ascolto della persona offesa entro tre giorni dalla denuncia. Le indagini terminano con una richiesta di archiviazione del procedimento, avverso la quale la denunciante propone opposizione, con udienza fissata al 10 dicembre prossimo. Aggiungo a tutto questo che, sempre secondo quanto si apprende dagli organi di stampa, la denunciante, in seguito alla denuncia sporta, avrebbe perso l'occasione di lavorare nella trasmissione "Piazza Pulita", in onda su LA7. Ora, tutti sappiamo quanto la corretta applicazione del codice rosso sia fondamentale per reprimere reati che destano un gravissimo allarme sociale. La disapplicazione di questa norma, che prevede un ascolto rapido della parte offesa, è quanto mai grave. pertanto al Ministro se intenda avvalersi dei propri poteri ispettivi per verificare la corretta applicazione dell'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, introdotto proprio dalla legge n. 69 del 2019.

commentare situazioni che sono in questo momento sotto l'indagine autonoma e indipendente della magistratura.

prevede effettivamente che entro tre giorni debba essere ascoltata la parte offesa, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della parte offesa. Quindi, nei limiti del rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, noi ci siamo attivati per chiedere alla procura di Roma una relazione informativa su questo. Nella serata di ieri è pervenuta la nota di trasmissione a firma del procuratore aggiunto della relazione informativa, che era stata firmata dal sostituto procuratore assegnatario del fascicolo, con allegato il decreto di differimento dell'audizione della persona offesa del 3 febbraio 2023 (come ho detto prima, può essere differita l'audizione della parte offesa) e la richiesta di archiviazione datata luglio 2023.

Quindi, nel decreto non risultano esplicitate le ragioni di questo differimento. Di conseguenza, è stata

a seguito di integrazione di istruttoria da parte dei nostri uffici, il procuratore della Repubblica di Roma ha trasmesso una "nota di chiarimento" a firma del pm titolare delle indagini, che, a integrazione della precedente relazione che ho indicato prima, testualmente recita «non si è ritenuto di dover assumere a sommarie informazioni la parte offesa all'esito della effettuazione delle attività di indagine prontamente avviate e prima del deposito della richiesta di archiviazione risiede nel fatto che, come già evidenziato in precedenza, la denuncia querela è stata raccolta da ufficiali di polizia giudiziaria specializzati nella materia dei reati contro la libertà personale, con proposizione di domande anche di approfondimento alla parte offesa in relazione al suo narrato, sicché la sua audizione, oltre a rivelarsi superflua, poteva aumentare il rischio di vittimizzazione secondaria». Da ex magistrato, posso dire che, effettivamente, la denuncia della parte offesa non equivale all'audizione della parte offesa nel termine dei tre giorni. Del resto, non è dato evincere dagli atti che sono stati trasmessi la delega del PM procedente alla Polizia giudiziaria per l'audizione entro il termine previsto dalla legge. Sulla scorta di queste risultanze, saranno interessate le articolazioni ministeriali per gli opportuni approfondimenti e le valutazioni di competenza. PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Campione, signor Ministro, mi dichiaro soddisfatta della sua risposta. Lei ha la nostra più completa fiducia nelle misure e negli accertamenti che vorrà disporre e le misure che vorrà adottare. Tutti sappiamo quanto sia importante la corretta applicazione del codice rosso per arginare le violenze di cui quotidianamente veniamo a conoscenza e questo è tanto più importante se teniamo conto che di recente è stata approvata una legge, che prevede addirittura che, in caso di mancato ascolto da parte del pm della persona offesa, si possa procedere addirittura all'avocazione delle indagini. Questo proprio a sottolineare quanto sia importante la tempestività nell'ascolto di chi le violenze, purtroppo, le subisce. *(Applausi)*.

mi sembrava giusto omaggiare anche in quest'Aula i novant'anni anni di una grande attrice italiana e una grande donna, Sophia Loren, al secolo Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, nata il 20 settembre del 1934 a Roma. Domani festeggerà il compleanno in una festa privata in cui si rivedrà il film che l'ha resa famosa come pizzaiola «L'oro di Napoli», film del regista Vittorio De Sica, con cui poi ha girato altri film. «È stata la prima volta della mia vita» - ha detto Sophia Loren - «che qualcuno ha creduto in me e ha scommesso su di me, non lo dimenticherò mai». Qualche giorno fa, in un'intervista a «la Repubblica» di Natalia Aspesi, che le chiedeva quale dei suoi tantissimi film lei metterebbe in un santuario, al massimo due, lei risponde: lei risponde: «"La ciociara" e "Una giornata particolare". Sì, metterei quelli. Sono due film di cui sono estremamente orgogliosa, perché rappresentano nel senso più profondo il mio lavoro come attrice. Sono così orgogliosa dei momenti che ho creato in questi film, insieme ai registi naturalmente, momenti che hanno toccato i cuori delle persone in tutto il mondo ma che hanno anche parlato alle donne in modo molto diretto. Non posso però non aggiungere a questa risposta anche il mio ultimo film, "La vita davanti a sé"». a sé"». Se con De Sica che la dirige diventa la pizzaiola d'Italia, un'icona a vita, l'attrice ha dovuto però imporsi, lottare come tante altre donne per la sua passione, scegliere di non tornare a Pozzuoli, dove viveva con la madre, per seguire il suo desiderio di diventare attrice. Ha vissuto, come tutte le altre donne, le lotte per il lavoro, l'indipendenza e contro la guerra. Con «La ciociara» vince l'Oscar, dato per la prima volta a un'attrice non di lingua inglese che rappresentava le speranze di una generazione uscita dal fascismo. Era così inedito che lei non credeva di poter battere Audrey Hepburn in «Colazione da Tiffany» e rimase a Roma. Il 9 aprile 1962 ricevette la telefonata che l'avvisava dell'Oscar. In «Una giornata particolare», capolavoro di Scola, conosce in un casermone, i palazzi Federici qui al quartiere Nomentano, mentre Mussolini e Hitler si stringono la mano il 6 maggio 1938, un gentile inquilino, abile nei passi di danza - è Mastroianni, con cui poi ha girato dodici ma prossimo al confino perché omosessuale. In fondo anche lei è una confinata, relegata alla vita domestica, un po' come Delia in «C'è ancora domani», il film della Cortellesi che, non a caso, Sofia Loren in questa intervista omaggia. Siamo però nel 1977 e questo è un film civile, pieno di umanità. Ancora, ne «La vita davanti a sé» - per stare solo a questi tre film - la Loren è una donna ex prostituta che accoglie un turbolento ragazzino di origine senegalese, piantando il seme di un profondo e reciproco affetto (a proposito di cittadinanza). È un film di cui lei è orgogliosa perché girato insieme al figlio. Sofia Loren è stata una grande diva ed ha ed ha interpretato film di successo con i più grandi registi: Monicelli, Scola, Dino Risi, Charlie Chaplin, Lumet. Tutti poi la ricordiamo per come nel 1999 consegna l'Oscar a Roberto Benigni, urlando «Roberto!». Una figura importante e straordinaria,